L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, anche considerata la diretta televisiva in corso. Il senatore Ferrazzi ha facoltà di illustrare l'interrogazione Interrogazione sul finanziamento dei progetti di rigenerazione urbana, in particolare rispetto alla quota assegnata ai Comuni del Nord Italia (**3-03007**)

Si tratta del finanziamento adeguato da garantire ai Comuni che hanno partecipato a un bando fondamentale, che tra l'altro è uno dei primi del PNRR, cofinanziato anche con questo fondo.

La differenza tra i progetti ammissibili e quelli che sono stati finanziati balza agli occhi. Per fare un esempio, nella mia Regione - il Veneto - sono stati finanziati solo 5 Comuni

che già il 70 per cento dell'inquinamento mondiale è nelle città. Questo vale anche nel nostro Paese. Quando parliamo di sviluppo delle città, parliamo dunque dello sviluppo del nostro Paese. È quindi importante che il Governo abbia contribuito in maniera determinante, attraverso capitoli di bilancio finanziati e rifinanziati, con un programma pluriennale fino al 2035. Signor Ministro, noi chiediamo che i 900 milioni di euro che mancano per finanziare tutti i progetti ammessi al bando vengano stanziati

come hanno ricordato gli onorevoli interroganti, la cornice giuridica di riferimento per l'erogazione dei contributi agli enti locali per investimenti in progetti di rigenerazione urbana ha trovato attuazione con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2021, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture, a seguito di un'intesa acquisita in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali con l'ANCI il 26 novembre 2020. In quella sede si è convenuto sulla necessità di introdurre, tra i criteri per la selezione dei progetti, quello che fa riferimento all'indice di vulnerabilità sociale e materiale definito dall'Istat. Si tratta di un criterio che trova applicazione quando, come nel caso in esame, l'entità delle richieste pervenute supera l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e che deriva dalla necessità di riconoscere una preferenza alle realtà locali più svantaggiate, in coerenza con la finalità dell'intervento legislativo. Pertanto, il decreto di individuazione dei Comuni risultati beneficiari è frutto dei criteri concertati in vista della distribuzione delle risorse. Appare evidente che la possibilità di erogare contributi anche in favore di progetti ritenuti ammissibili, ma che non hanno beneficiato delle risorse per l'incapienza dei fondi disponibili richiedeva un'ulteriore integrazione degli stanziamenti. Rammento che, dopo un primo intervento già effettuato con il decreto-legge n. 152 del 2021, che ha implementato nel quadro delle risorse del PNRR i fondi disponibili integrandoli di 200 milioni di euro per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, ulteriori interventi sono stati disposti con la legge di bilancio 2022 per corrispondere a queste esigenze di ampliamento della platea dei beneficiari. Si è stabilito che i fondi, integrati per il corrente esercizio di ulteriori 300 milioni, possono essere assegnati anche ai progetti presentati dai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che in forma associata superano detta soglia. Potranno concorrere a questo nuovo finanziamento anche quei Comuni che non sono risultati beneficiari del finanziamento proprio per insufficienza delle risorse. La legge di bilancio 2022 ha previsto che, a decorrere dal 2023, le Regioni potranno utilizzare le risorse già a esse assegnate per gli investimenti in tema di rigenerazione urbana, prevista dalla legge di bilancio 2019, proprio allo scopo di realizzare i progetti ricadenti nel proprio territorio ritenuti ammissibili. Tuttavia, ben consapevoli della delicatezza e della rilevanza della tematica e in coerenza con un apposito ordine del giorno approvato in sede di discussione della legge di bilancio 2022, assicuro che il Governo è impegnato nell'individuazione di ogni utile soluzione per andare incontro alle esigenze rappresentate in questa sede. ringrazio il Ministro per la risposta e soprattutto per il passaggio finale in cui si impegna a nome del Governo a trovare

sopra i 15.000 abitanti e non solo per le grandi città metropolitane o i Comuni capoluogo, ma anche per quei Comuni che spesso sono i piccoli motori del territorio, i riferimenti dei piani di zona e dei servizi locali e possono essere anche la vetrina con cui raccontiamo all'opinione pubblica e ai cittadini che il PNRR funziona, che c'è un ritorno sul territorio. Per ciò pensiamo davvero che sia importante affrontare non solo il tema, come giustamente facciamo nel PNRR, dei divari generazionali, di genere e tra Nord e Sud, dei divari all'interno delle stesse Regioni e delle stesse città. Un bando come questo serve anche ad affrontare quelle disparità che spesso vengono considerate secondarie. Consideriamo molto importante l'impegno che si è assunto. Sarebbe un segnale poter finanziare tutti i progetti che sono ammessi, per poter partire nella maniera migliore possibile.

considerato che il PNRR si sviluppa in sei missioni e riserva un finanziamento considerevole alla bonifica dei siti orfani, valutato che l'ufficio del commissario unico per le bonifiche ha rilevato due specifiche criticità circa la procedura di iscrizione in *white list* delle società di categoria X, che si occupano appunto di bonifiche e di servizi ambientali e, cioè, di casi di ditte la cui domanda di iscrizione rimasta non perfezionata e di ditte regolarmente iscritte, ma con richiesta di rinnovo dell'iscrizione pendente da anni; posto che per poter partecipare alle gare di appalto è considerata sufficiente la mera richiesta d'iscrizione e per l'aggiudicazione degli appalti pubblici la mera interrogazione della banca dati nazionale in una prefettura a elevata attività operativa come quella di Napoli il 12 ottobre 2021 su 1.076 società richiedenti inserimento in *white list* soltanto per 31 è indicato un esito, mentre le altre 1.045 risultano da anni in fase di valutazione e, pertanto, in attesa di iscrizione. Ben 139 su 1.045 domande riguardano la certificazione per la categoria X. Nel merito, poi, l'elenco delle citate 1.076 società conta 8 con richiesta di iscrizione per il 2014, 46 per il 2015, 118 per il 2016, 96 per il 2017, 144 per il 2018, 140 per il 2019, 172 per il 2020 e 352 (quindi più del doppio dell'anno precedente) per il 2021. Sempre a Napoli le società già iscritte, invece, sono in tutto 1.489, di cui 615 con richiesta di aggiornamento in iscrizione, 191 delle quali afferenti alla categoria X e solo 10 con diniego di iscrizione. Delle predette 615, 24 sono in attesa di aggiornamento dal 2016, 48 dal 2017, 54 dal 2018 e 64 dal 2019. Addirittura per 73 società, la cui iscrizione risulta scaduta, non sono neppure segnalati aggiornamenti in corso, pur permanendo le stesse nell'elenco. Signor Ministro, si chiede perciò di sapere se intenda verificare quale garanzia di indipendenza dalle infiltrazioni mafiose presentino le società inserite in *white list*, la cui verifica non risulta effettuata o rinvia ad un'istanza risalente nel tempo, e parimenti quali garanzie di efficienza garantisca l'interrogazione della banca dati nazionale antimafia (BDNA) prevista quale atto liberatorio per le aggiudicazioni di appalti pubblici. se, inoltre, intenda verificare quali siano le effettive motivazioni che non hanno reso possibile il perfezionamento di numerose posizioni di inserimento nelle *white list*, con speciale attenzione alle situazioni che risalgono ad oltre cinque anni da oggi e se il Ministro non reputi opportuno verificare la regolarità degli inserimenti e controlli in *white list* in tutte le prefetture d'Italia, anche alla luce della mancanza di uniformità della gestione e presentazione dei dati degli elenchi da parte dei suddetti uffici di Governo, al fine di garantire un agevole utilizzo dello strumento da parte delle stazioni appaltanti e l'effettiva validità delle procedure previste per l'esclusione delle società da infiltrazioni mafiose. PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, consigliere di Stato Lamorgese, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, Signor Presidente, è opportuno precisare che il sistema della documentazione amministrativa è stato concepito dal legislatore per garantire le necessarie verifiche, senza tuttavia paralizzare l'attività imprenditoriale. Infatti il codice antimafia prevede che, qualora le verifiche esperite non si concludano nei tempi prescritti, le pubbliche amministrazioni possono procedere anche in assenza delle informazioni antimafia, fermo restando che in caso di esito negativo degli accertamenti sarà disposta necessariamente la revoca dei provvedimenti ampliativi, ovvero attivato il recesso dai contratti. Per quanto riguarda le criticità evocate in merito ai tempi di iscrizione nelle *white list*, occorre porre in luce che la relativa attività istruttoria è condizionata da molteplici fattori, relativi al contesto territoriale di riferimento e alla complessità degli accertamenti che a volte possono richiedere l'interessamento di varie prefetture. Per quanto riguarda la specifica situazione di Napoli, è evidente come sui tempi di evasione delle richieste di iscrizione nelle *white list* incidano significativamente fattori di criticità legati a quel contesto territoriale, ciò sia per l'elevato numero delle istanze, sia per la complessità delle dinamiche criminali, la cui analisi finisce per condizionare la definizione delle singole posizioni. Il prefetto di Napoli ha precisato anche che tra i vari fattori che concorrono a prolungare la durata del procedimento istruttorio, il più frequente è rappresentato dalle variazioni degli assetti societari o delle composizioni familiari, che implicano ogni volta l'avvio di nuovi accertamenti. Peraltro, periodicamente la prefettura di Napoli provvede a verificare la persistenza dell'interesse delle società all'iscrizione nelle *white list*, allo scopo di snellire i carichi di lavoro da un lato e di concentrare gli accertamenti sulle istanze per le quali si riscontri invece l'attualità dell'interesse. È doveroso anche precisare che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 76 del 2020, le informazioni antimafia e le iscrizioni in *white list* ricevono la stessa disciplina: laddove non sia possibile rispettare i tempi di rilascio, sono comunque precedute

si dà corso al rilascio dell'informativa liberatoria provvisoria, che consente di accedere ai contratti pubblici sotto condizione risolutiva, destinata a operare quando gli ulteriori accertamenti si concludano negativamente. Tengo infine a precisare che il Ministero dell'interno lo scorso 13 dicembre ha diramato una circolare ai prefetti con cui, nel sottolineare l'attuale contesto storico caratterizzato dalla necessità di dare sollecita attuazione agli obiettivi del PNRR, è stato richiesto un particolare impegno per contenere al massimo i tempi di trattazione delle pratiche di iscrizione nelle *white* *list*, al fine di creare i presupposti per una ripresa economica in piena trasparenza, il più possibile scevra da rischi di infiltrazione criminale.

personale delle prefetture che si impegna in queste attività. Dal momento che a me non risulta ci sia del personale dedicato, ho l'impressione che sul territorio ciascuna prefettura agisca sulla base delle proprie possibilità. Da

non c'è un monitoraggio, non esiste e non è possibile perché, come ho detto nell'illustrazione, ogni prefettura addirittura adotta un proprio criterio nello stendere gli elenchi. Ce ne sono alcune che, ad esempio, non riportano neppure la categoria per la quale la singola società fa domanda. quindi una certa discrezionalità che poi va a ripercuotersi sulla possibilità di avere un quadro e di monitorare la situazione.

Signor Presidente, signora Ministro, come purtroppo sappiamo a Milano, nella notte di Capodanno, almeno nove giovani donne sono state vittime di molestie e violenza sessuale. Come possiamo vedere sui numerosi video che circolano in rete e secondo quanto riportato dagli organi di informazione, 18 ragazzi, 15 maggiorenni e tre minorenni, tra i quindici e i sia stranieri che italiani di origine nordafricana di seconda generazione, sono stati identificati perché ritenuti coinvolti nelle aggressioni a sfondo sessuale. Secondo quanto risulterebbe dagli accertamenti degli inquirenti vi sarebbero almeno tre diversi episodi di violenza consumati sempre a Milano in piazza Duomo nella notte di Capodanno. Questi tre episodi vedono coinvolti questo gruppo di giovani e giovanissimi che sembrano agire in branco, ma soprattutto in maniera organizzata.

centinaia di stranieri e cittadini tedeschi di origine nordafricana si sono avventati contro donne intente a festeggiare il Capodanno, provocando vere e proprie azioni di guerriglia organizzata, finalizzate ad aggressioni sessuali. Sappiamo ovviamente che la violenza contro le donne è un problema che riguarda tutte le società, ma va posta l'attenzione sulla pervasività di talune culture che hanno nel tempo radicalizzato una visione della donna fortemente discriminatoria, posta in condizione di subalternità e in netto contrasto con i principi della nostra Costituzione che si fondono sulla cultura democratica che da millenni appartiene all'Occidente. Preoccupa il fatto che in alcuni Paesi arabi della regione nordafricana la molestia collettiva su una donna sia una pratica che ha avuto un incremento esponenziale negli ultimi vent'anni, seguendo il percorso di radicalizzazione religiosa. Vi sono aree e quartieri privi di qualsiasi forma di controllo, specialmente negli Stati europei dove c'è un maggior tasso di immigrazione. Questo può comportare il rischio di un aumento dei fenomeni come quelli descritti ed evidenzia l'incapacità di prevedere stabili processi di integrazione. Preoccupa la non gestione del fenomeno, soprattutto negli Stati membri ad alta densità migratoria e c'è una grande difficoltà nel contrastare il proliferare di questi gruppi di giovanissimi, che non riconoscono i sistemi valoriali dei nostri Paesi europei.

nell'esprimere la mia solidarietà alle vittime di tali gravissime aggressioni, desidero preliminarmente informare in merito alle iniziative finora svolte per individuare i responsabili e assicurarli alla giustizia. Evidenzio, innanzitutto, che la presenza di personale della questura di Milano nel luogo in cui sono accaduti i fatti ha consentito, per il più grave degli episodi, di intervenire tempestivamente, mettendo in fuga gli aggressori. Sui fatti in questione, la squadra mobile di Milano, di concerto con l'autorità giudiziaria, ha immediatamente attivato capillari analisi per l'identificazione dei responsabili, anche mediante ricorso a fonti aperte e *social network*, procedendo all'acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. Nel quadro delle indagini così disposte sono state eseguite perquisizioni domiciliari e personali a Milano, Torino e Bergamo nei confronti di 18 soggetti, di cui tre minorenni, sia di nazionalità italiana che straniera. All'esito di tale attività investigativa, il pubblico ministero ha eseguito il decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di due soggetti ritenuti responsabili del delitto di violenza sessuale. Nei confronti degli stessi, il questore di Milano ha adottato il provvedimento del foglio di via obbligatorio e dell'avviso orale. Ribadisco che quelli di Milano sono fatti gravissimi ed inaccettabili e assicuro che le Forze di polizia profonderanno il massimo impegno per garantire la sicurezza delle nostre città per evitare che possano ripetersi analoghi comportamenti, anche tramite un eventuale adeguamento dell'organico ivi presente. Riguardo ai profili richiamati dall'interrogante, relativi al rispetto della figura femminile e alla ripulsa per ogni spregevole comportamento offensivo della libertà e della dignità della donna, specie se commesso con la complicità del vile anonimato del branco, condivido la necessità, rappresentata dall'onorevole interrogante, di una profonda azione di intervento sociale in chiave educativa e preventiva. La risposta dello Stato e delle istituzioni non può limitarsi, infatti, alla sola, pur essenziale, componente repressiva. Occorre sviluppare appropriate politiche di riduzione del disagio sociale, maggiormente nelle fasce della popolazione giovanile e negli ambiti urbani esposti a fenomeni di degrado e devianza. L'obiettivo è quello di evitare qualunque forma di ghettizzazione che faccia da collante al risentimento e all'odio sociale e che finisca con il risultare antitetica rispetto all'esigenza di un'effettiva integrazione comunitaria. potrò dirmi soddisfatta quando vedrò nei fatti *(Applausi)* che ci sarà un cambiamento radicale nella gestione del fenomeno migratorio. Se è vero che c'è il grosso problema della redistribuzione, sappiamo che noi - dobbiamo pensare al nostro Paese, ognuno penserà al suo - possiamo agire veramente facendo quanto ha appena detto su numeri limitati, perché maggiori saranno gli arrivi di massa più sarà difficile gestire l'integrazione. Lo dico anche da sindaco di un piccolo Comune dove gli immigrati non sono considerati stranieri, ma hanno un nome, un cognome, un volto; ma non si può continuare a lasciare tutto il peso dell'integrazione sulle scuole, soprattutto in questo periodo in cui i giovani hanno già tanti problemi dovuti alla pandemia, alla DAD e a quanto ne consegue. Non si può lasciare tutto il peso dell'integrazione sui Comuni o sul volontariato. Quando arrivano sul nostro territorio,

ma so perfettamente che ci sono enormi problemi di scontri culturali, e se in casa la famiglia di prima generazione che non ha avuto un'integrazione dà insegnamenti non in linea con i nostri valori, ovviamente il ragazzo non capirà mai quale sia la linea giusta da seguire: a scuola gli si insegna una cosa, a casa gliene insegnano magari un'altra (non tutti, perché ci sono anche famiglie integrate). Quindi, bisogna agire in fretta perché questi episodi sono la punta di un iceberg. Anche nei nostri piccoli centri si notano fenomeni preoccupanti

finestra") *(M5S)*. Ministra Lamorgese, negli ultimi giorni si sono susseguiti numerosi attentati dinamitardi nei confronti di attività economiche a San Severo e a Foggia. Un numero così alto di bombe, racchiuse in un lasso di tempo così breve, ha destato grande preoccupazione, sgomento e allarme tra i cittadini, e purtroppo questi attentati non costituiscono una novità nel nostro territorio, visto che nei mesi e negli anni scorsi abbiamo dovuto registrare molti accadimenti analoghi a danno di altre attività economiche, ma anche a danno delle Forze dell'ordine. Solo per fare qualche esempio, ricordo a San Severo colpi di arma da fuoco nei confronti di un automezzo della Polizia di stato; a Cerignola un ordigno devastò l'autovettura del comandante della locale stazione dei Carabinieri oppure atto ai danni di un sottufficiale sempre dell'Arma a Corato o addirittura la bomba fatta esplodere davanti al commissariato di Canosa di Puglia. Queste modalità cruente ed eclatanti utilizzate dalle compagini mafiose hanno il palese obiettivo di intimidire e di prostrare la cittadinanza e gli operatori economici al fine di portare a termine gli obiettivi criminali. D'altro canto, lo Stato - occorre sottolinearlo - specie in questi ultimi quattro anni, ha conseguito successi importantissimi procedendo a centinaia di operazioni antimafia, centinaia di arresti che hanno portato in carcere, a scontare condanne passate in giudicato o in attesa di sentenze definitive,

e ben cinque gli scioglimenti di Consigli comunali, compresi quelli del Comune capoluogo. Tutto ciò grazie al coraggio e alla professionalità di uomini e donne della magistratura, delle Forze dell'ordine e delle diramazioni governative territoriali. Evidentemente, però, tutto ciò non è sufficiente. Bisogna fare ancora di più per controllare maggiormente il territorio e per difendere i cittadini. Le importanti città di San Severo e Cerignola, con i loro 60.000 abitanti, che, come detto, sono interessati da pericolosi *clan* mafiosi, non sono dotate di commissariati della Polizia di Stato di cosiddetto primo livello, con tutto ciò che ne consegue in termini di minori risorse tecniche e umane e capacità investigative. Crediamo sia necessario incrementare il numero di poliziotti in queste due città, quindi elevare urgentemente i suddetti commissariati a strutture di primo livello, e a tal fine

foggiane, perpetrata a danno di esercizi commerciali locali, che ha destato particolare allarme sociale. È noto come il contesto foggiano risulti da tempo caratterizzato da una significativa evoluzione della criminalità organizzata locale, la quale, in analogia al *modus operandi* di altre consorterie mafiose, ha orientato i propri interessi verso il tessuto economico e sociale e quello amministrativo, col chiaro intento di infiltrarsi in tali ambiti per il perseguimento dei propri fini illeciti. La reazione dello Stato, tuttavia, non è mancata, come testimoniano l'attività svolta dalla magistratura e dalle Forze di polizia, intensificatasi dopo l'eccidio di San Marco in Lamis del 2017, e anche la recente istituzione, nel febbraio 2020, di una sezione operativa della DIA con sede proprio a Foggia. Sono stati raggiunti anche in questi anni significativi risultati sul piano dell'azione repressiva, con l'adozione - come ricordato dall'onorevole interrogante - di circa 400 misure cautelari, il sequestro di ingenti quantitativi di droga, di armi, munizioni e ingenti patrimoni, per un ammontare complessivo Parallelamente, sul versante della prevenzione antimafia, sono state adottate 67 interdittive a carico di imprese collegate o condizionate dalla criminalità organizzata foggiana, mentre l'azione di vigilanza sui tentativi di infiltrazione nelle amministrazioni locali ha portato recentemente allo scioglimento del Consiglio comunale di Foggia, che fa seguito ad altri scioglimenti, quali quelli di Mattinata, Cerignola e Manfredonia. Non c'è dubbio che l'innalzarsi dell'offensiva mafiosa, in particolare nel comune di San Severo, determini la necessità di un'ulteriore intensificazione dell'azione di prevenzione e contrasto, proprio per riaffermare i principi di legalità e ripristinare i livelli di sicurezza

a cui parteciperanno anche i vertici delle Forze di polizia, il capo della Polizia, i comandanti generali della Finanza e dei Carabinieri, e in più i vertici nazionali della magistratura antimafia. Alla riunione parteciperà anche il Commissario antiracket e antiusura, proprio in considerazione del fatto che, in quella stessa giornata, verrà presentata un'associazione antimafia e antiusura intestata proprio alla memoria dei fratelli Luciani, vittime dell'agguato di San Marco in Lamis. In sede di comitato sarà operata una valutazione delle misure che dovranno essere assunte e la mia visita a Foggia sarà anche l'occasione per un confronto con il sindaco e gli amministratori del Comune di San Severo, per fare un punto di situazione. Vorrei però dare anche dei dati più precisi che riguardano la questione degli organici delle Forze di polizia. Informo che tra il 2020 e il 2021 il personale della Guardia di finanza è stato rafforzato

Quindi, sta di fatto che, anche in base al piano di ridefinizione e riassetto organico, messo a punto dal Dipartimento della pubblica sicurezza a livello nazionale, ma anche a livello territoriale, ulteriori 50 operatori saranno progressivamente assegnati alla questura di Foggia, che pertanto, al compimento di questo programma di ampliamento e rafforzamento, passerà dalle attuali 497 a 547 unità.

delle Forze dell'ordine. Dobbiamo rimarcare la situazione e voglio riferire le parole del Procuratore nazionale antimafia, che è l'esponente principale del contrasto alle mafie nel nostro Paese, il dottor Cafiero De Raho, che in più di un'occasione ha parlato della situazione mafiosa di Foggia come di un'emergenza nazionale. Quindi, se l'attuale situazione costituisce un'emergenza, occorre avere il coraggio e la forza - che non le mancano, signora Ministra

Confidiamo nella sua azione: ha già dato dimostrazione, nei primi mesi della sua nomina a Ministra nel Governo precedente, di saper agire immediatamente, quando approvò

Signor Presidente, signor Ministro, visto che il Ministero è impegnato correttamente nella realizzazione di importanti infrastrutture, a maggior ragione oggi, con il Piano nazionale di ripresa e resilienza e con i grossi investimenti che saranno realizzati proprio in ambito infrastrutturale, un'opera lunga 140 metri e larga 30 metri rischia di essere assolutamente sottovalutata, se non se ne comprende la portata. Il ponte Corleone, che è tanto piccolo, è tanto strategico per la città di Palermo, perché questo ponte e la circonvallazione sono l'unica strada che consente il passaggio

all'interno della città stessa. Se quest'opera continua a essere sottovalutata per quanto riguarda l'importanza della sua realizzazione, rischiamo di continuare a far vivere un grossissimo disagio alla quinta città d'Italia. È un ponte che non è stato messo in sicurezza, che era stato finanziato e di cui si sono perse le risorse. Con un emendamento di Italia Viva abbiamo richiesto il commissariamento di quest'opera, proprio per l'incapacità del Comune di Palermo di trovare una soluzione e di risolvere il problema. Ancora oggi ci sono difficoltà: crediamo ad esempio che il cronoprogramma di intervento su quest'opera debba prevedere inizialmente la realizzazione delle due corsie laterali, in modo da mettere in sicurezza successivamente il ponte ed evitare che ci sia una situazione di blocco totale della città. Noi le chiediamo, signor Ministro, di dare la giusta importanza alla realizzazione di questa infrastruttura, che è fondamentale per la mobilità della quinta città d'Italia. Questo *question time* è l'opportunità per ascoltare che cosa vuole mettere in campo il Ministero, oltre al commissariamento, al fine di consentire alla città di Palermo di vedere finalmente realizzato questo intervento.

è stato stipulato uno specifico protocollo d'intesa tra il Comune di Palermo, il provveditorato interregionale per le opere pubbliche Sicilia e Calabria e l'ANAS. A tale protocollo d'intesa ha fatto seguito la convenzione attuativa dell'intervento, denominata «Risanamento della struttura in cemento armato e interventi da realizzare sul ponte Corleone», sottoscritta in data 5 luglio 2021, con la quale ANAS ha assunto il ruolo di stazione appaltante. Condividendo l'importanza cruciale di questa opera e al fine di accelerare la realizzazione degli interventi - come lei ha ricordato - si è proceduto alla nomina di un commissario straordinario, con il compito di procedere, tra l'altro, al risanamento della struttura in cemento armato, alla realizzazione degli ulteriori interventi necessari, alla costruzione dei ponti laterali sul fiume Oreto al completamento dei lavori di costruzione del raddoppio della circonvallazione di Palermo da via Altofonte a via Belgio. Riguardo al primo intervento, il 4 gennaio - qualche giorno fa - si sono concluse le indagini, comprese le prove di carico dinamiche e l'analisi di sicurezza sarà rilasciata entro il 15 febbraio 2022. Per il secondo intervento sono attualmente in corso le indagini integrative sulle opere a suo tempo parzialmente eseguite e la redazione del progetto definitivo delle nuove opere, che è necessario per l'avvio delle procedure approvative e la convocazione della relativa conferenza dei servizi. Quanto al terzo intervento, è in corso un'interlocuzione tra il commissario straordinario e gli uffici del Comune di Palermo per valutare l'ipotesi di ricorrere a un apposito accordo quadro, volto a superare le criticità finora riscontrate. Considerata l'indubbia strategicità dell'opera come collegamento tra la A29 e la A19 e per la viabilità locale, il Ministero, attraverso la società ANAS, ha già cercato di accelerare il processo e continuerà a svolgere questi approfondimenti. Nei giorni scorsi ho trasmesso alle Camere il rapporto sull'esito dei commissariamenti e quindi i cronoprogrammi e proprio oggi abbiamo concordato con il Vice Ministro competente per gli interventi stradali un intervento specifico per singola opera, in particolare per il ponte Corleone, per vedere come accelerare il cronoprogramma fornito dai commissari.

Ministro, se in questo momento lei dovesse transitare da Catania verso Palermo-Punta Raisi, troverebbe file infinite di persone incolonnate costantemente giorno per giorno su un'opera che, lo ripeto, non ha alternative.

a mia prima firma, se intende adoperarsi per porre rimedio a una criticità grave del settore ferroviario privato e dei trasporti su gomma a media e a lunga

proposta di interrogazione, qualcosa si è mosso - sono abbastanza informato - ma voglio essere certo che un pacchetto di misure che comprenda ad esempio il prolungamento della cassa integrazione, ma anche tutti i sostegni possibili alle aziende che operano in regime di concorrenza libera e privata, possa essere dato: penso all'abbattimento dei pedaggi sia autostradali sia ferroviari; penso a tutta una serie di ristori che possono e debbono essere dati, perché il settore coinvolge direttamente i cittadini, ma anche tanti lavoratori, tante imprese e tante attività industriali che fanno parte della ricchezza del nostro Paese.

Signor Presidente, la pandemia da Covid-19 e le conseguenti politiche di regolamentazione e limitazione degli spostamenti hanno modificato le tendenze di mobilità dei cittadini e delle merci, anche se va evidenziato come l'attuale fase emergenziale rappresenti un quadro certamente più positivo della situazione iniziale, che aveva portato al *lockdown* di molte attività. Per far fronte ai danni causati dall'emergenza Covid-19 sono state stanziate significative risorse, pari a circa otto miliardi di euro, destinate al settore del trasporto ferroviario, su gomma, marittimo e aereo, cui si aggiungono quelle finalizzate al finanziamento della cassa integrazione, alla moratoria dei pagamenti anche tributari e delle altre misure di sostegno agli investimenti, in particolare delle piccole e medie imprese. Ricordo anche che il trasporto pubblico locale è stato oggetto di un intervento molto forte, con uno stanziamento complessivo di 2,7 miliardi di euro, di cui 1,2 miliardi negli ultimi dieci mesi (tutti già ripartiti ed erogati). Segnalo, da questo punto di vista, che il Governo aveva stanziato 840 milioni per i servizi aggiuntivi nel secondo semestre del e che, a fronte del fatto che, nonostante le nostre indicazioni, le Regioni che hanno la responsabilità del trasporto pubblico locale hanno ritenuto di non usare tutti i fondi a loro disposizione, c'è la possibilità di usare i residui anche per coprire le perdite (mi riferisco al trasporto pubblico locale). Mi dispiace, senatore La Russa, ma noi già dalla scorsa settimana abbiamo iniziato a lavorare proprio in preparazione del prossimo decreto-legge annunciato dal Presidente del Consiglio, e sulla base delle prime evidenze nell'ultimo bimestre c'è un significativo decremento dell'attività di trasporto, come lei ha ricordato. Proprio in considerazione di tale contrazione, il Ministero sta definendo il nuovo quadro esigenziale, che, in linea con quanto già previsto nei precedenti provvedimenti d'urgenza, riguarda l'intero settore dei trasporti, individuando, in stretto coordinamento con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse occorrenti a tal fine. Come lei ha ricordato, proprio durante questa settimana ci sono stati incontri per definire questo quadro esigenziale.

che ci sono quell'emergenza e quell'esigenza che le rappresento. Quando mi dice che già da qualche giorno ci state pensando, non fa altro che confermare il motivo della nostra interrogazione urgente, e cioè che c'è bisogno che, oltre a pensarci, vi decidiate a realizzare concretamente un aiuto, non solo snocciolando cifre più o meno

del trasporto su gomma a media e lunga distanza - bensì anche per i cittadini. La conseguenza sarebbe un disservizio sui trasporti, se dovessero chiudere, che ricadrebbe sulla possibilità dei cittadini di usufruire di servizi che i privati forniscono in aiuto ai servizi pubblici. Mi dichiaro pertanto in attesa di poter essere soddisfatto, ma è un'attesa vigile, perché continueremo a verificare che, al di là delle parole, arrivino i fatti, esattamente come facciamo per il sistema del turismo, degli impianti sportivi, del *food*, del divertimento e di altri settori che stiamo controllando. Voi vogliate non a parole, ma nei fatti, cercare di aiutare.

per portare all'attenzione del Governo, che ha recepito (e ringrazio il Ministro per il lavoro svolto fino a oggi),

tra il Lazio e la Liguria, che impedisce un transito in totale sicurezza, come avviene in altre parti del territorio. Spesso ricordo che anche noi abbiamo l'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Si parla sempre di quella da prima che nascessi e spero che non si continuerà a parlare dell'asse della tirrenica ancora dopo che non saremo più in questo benedetto mondo.

l'attività del Ministero che lei presiede. Lo abbiamo fatto anche per rendere noto alla comunità che ci ascolta l'impegno che il Governo e la maggioranza stanno mettendo in questa direzione. Vorremmo sapere formalmente da lei, che presiede il Dicastero, le date per quanto riguarda la progettazione e la realizzazione della variante Aurelia tirrenica e dell'alta velocità. Le rivolgo inoltre una preghiera. Nel frattempo, per dare dignità ai passeggeri che oggi utilizzano la rete ferroviaria italiana anche nel tratto della strada Tirrenica, mandiamo in pensione i vecchi pendolini e piazziamoci un ETR1000, che andrà sicuramente a media-bassa velocità, ma almeno offrirà dignità e qualità per un trasporto moderno che l'Italia già porta avanti in altre realtà del territorio. PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, professor Giovannini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre con riferimento all'oggetto della richiesta dei senatori interroganti, confermo la grande attenzione posta dal Governo sullo sviluppo delle interconnessioni autostradali e ferroviarie che riguardano il versante tirrenico della nostra penisola. In attuazione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 e in ottemperanza alle decisioni assunte dalla Corte di giustizia europea, il Ministero sta procedendo alla revisione del rapporto concessorio con il concessionario, Società Autostrada Tirrenica (SAT). Al fine di assicurare il riequilibrio delle condizioni economico-finanziarie e accelerare la sottoscrizione della nuova convenzione, la legge di bilancio per l'anno 2022 ha previsto l'erogazione di un contributo pubblico pari a complessivi 200 milioni di euro per il periodo 2022-2026. Ai fini del riconoscimento di detto contributo, la società SAT è tenuta a presentare, entro il termine del 31 gennaio 2022 (quindi tra qualche settimana) un piano economico-finanziario predisposto in conformità alla disciplina regolatoria definita dall'Autorità di regolazione dei trasporti. Quanto all'entità del contributo da riconoscere effettivamente alla società concessionaria, è stato previsto che la stessa venga determinata all'esito della verifica da parte del Ministero, nell'ambito della valutazione della proposta di piano economico-finanziario presentata dalla predetta società, del raggiungimento delle condizioni di equilibrio e sostenibilità tariffaria della concessione. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dell'intervento viario Tarquinio-San Pietro in Palazzi è stato inoltre autorizzato l'acquisto da parte della società ANAS dei progetti elaborati dalla SAT relativi al predetto intervento, stanziando a tal fine l'importo di 36,5 milioni di euro. Inoltre, è stata prevista l'assunzione da parte dell'amministratore delegato di ANAS nel ruolo di commissario straordinario, in modo tale da poter procedere speditamente ai lavori. Quanto al progetto della ferrovia tirrenica, rappresento che RFI ha in corso interventi di potenziamento prestazionale tra La Spezia e Genova, nonché di rinnovo delle tecnologie sull'intero itinerario tirrenico tra Genova e Roma. Inoltre, RFI ha comunicato l'intenzione di svolgere specifici studi di fattibilità finalizzati alla verifica della possibilità di procedere alla velocizzazione di alcune tratte di detta linea. In questo modo, all'interno del contratto di programma di RFI sarà possibile stanziare i fondi. Infine, quanto ai collegamenti tra Genova, Pisa e Roma via Firenze, RFI ha comunicato che sono in corso interventi di velocizzazione nelle tratte comprese tra Pisa e Firenze, che consentiranno di ottenere consistente riduzioni del tempo di viaggio. Evidentemente, per ciò che riguarda il materiale rotabile, i treni modelli ETR 1000 per caratteristiche costruttive e prestazionali sono destinati a un utilizzo su linee di alta velocità esistenti. Ciononostante, valuteremo la possibilità di proporre a Trenitalia l'utilizzo di questi treni anche sulla linea tirrenica. Presidente, Ministro, sull'ultima questione degli ETR1000 l'anno scorso, grazie a una richiesta del sottoscritto, è stato fatto un esperimento. Nel periodo estivo sono stati messi due ETR

La funzionalità è sicuramente garantita; bisogna vedere se c'è un po' di volontà da parte di RFI. Sono soddisfatto degli acquisti dei progetti di SAT da parte di ANAS e questo è estremamente importante.

L'altra questione è l'attenzione estrema al 31 gennaio per la presentazione da parte di SAT. Stiamo tutti aspettando questo momento per chiudere la partita dei 200 milioni. Ringraziandola e ritenendomi estremamente soddisfatto della risposta che oggi ci ha fornito e riprendendo una questione legata a quanto si diceva prima sui ristori per le imprese e sui trasporti, ricordo che è ancora sospeso quel ristoro da 50 milioni per i bus turistici dello scorso anno e non è ancora uscito il bando. La inviterei quindi, nelle more della sua disponibilità, che è sempre massima e totale, a farci mettere un po' di attenzione dagli uffici, perché le imprese dei bus turistici, che hanno sofferto così tanto,